L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

decise da organismi sovranazionali, alle quali l'Italia partecipa con contributi molto significativi. Non sono solo una parte importante della politica estera del nostro Paese, ma proprio la maniera in cui oggi si concepisce - queste sono le nuove sfide le nuove sfide della sicurezza - il modo di gestire la sicurezza del Paese: queste sono le minacce attuali, nuove, e questo è il modo di rispondervi. Proprio per questo motivo è corretto ed importante che oggi in quest'Aula,

...sono state assunte decisioni importanti, soprattutto nell'ambito delle risorse assegnate, che credo necessitino di una riflessione più ampia di quella fatta in Commissione. Facciamo un passo indietro.

nel corso di un certo numero di anni e sulla base di aggiustamenti progressivi. Il modello a 190.000 unità prevede 22.000 ufficiali, 64.000 sottufficiali, 104.000 unità di truppa.

cambia radicalmente nel momento in cui si decide di passare ad un modello professionale. Da un lato, la politica chiede alle Forze armate di anticipare e velocizzare una trasformazione assolutamente necessaria,

ma nel 2010 è previsto un taglio del reclutamento del 40 per cento. Se rimane questo stato di cose,

gravissimo, sentito in modo molto profondo da chi opera nelle nostre Forze armate. In merito, c'è una preoccupazione causata dall'ipotesi

Nel settore dell'esercizio, rispetto al 2008, vi è un decremento di 775 milioni di euro (circa il 29 per cento) e i volumi finanziari risultano assolutamente insufficienti per assicurare, sia pure al minimo livello di adeguatezza, le attività di addestramento e di formazione, le attività di manutenzione e le scorte di materiali,

(lo abbiamo già ricordato, ma voglio farlo anche qui): il Capo di Stato maggiore della Difesa, sentito nelle Commissioni difesa di Camera e Senato, ha lanciato un allarme pesantissimo, in sede parlamentare che c'è il rischio di un progressivo decadimento operativo dello strumento militare, a seguito di una riduzione, prossima all'azzeramento, delle esercitazioni, delle ore di moto e di volo delle varie componenti e della sensibile

con il compito di dare un riassetto alle Forze armate e procedere a una revisione del modello di difesa esistente. Non c'è nessun problema a riconoscere l'esigenza di razionalizzare,

una Nazione che confina con noi ha appena lavorato per definire un modello di difesa, e mi riferisco alla Francia. Come ha lavorato su questo Libro bianco? Ha messo in piedi una commissione che intanto

Ha facoltà di parlare il senatore Galioto per illustrare la mozione n. 147. è caratterizzato da molteplici situazioni di criticità, derivanti soprattutto dall'accentuazione dei processi di frammentazione e di instabilità, dall'aggravamento e dall'esplosione, sotto molteplici forme, dei fenomeni terroristici e di criminalità transnazionale, ma anche dalla grave crisi finanziaria ed economica che potrebbe influenzare negativamente nei prossimi mesi l'evoluzione degli scenari di crisi. La presenza di realtà statuali deboli e disgregate e lo sviluppo di reti terroristiche in grado di estendere le proprie aree di reclutamento ed addestramento costituiscono le principali minacce per la sicurezza e la stabilità mondiale. Contestualmente la proliferazione delle tecnologie e delle capacità associate alle armi di distruzione di massa provoca effetti destabilizzanti che vanno anche oltre l'utilizzo stesso di questi sistemi. Questi scenari e l'eterogeneità delle crisi che si sviluppano nelle varie parti del mondo, pertanto, implicano un'estensione del tradizionale concetto di difesa volto soprattutto alla tutela e alla salvaguardia degli interessi nazionali, richiedendo un approccio più ampio alla sicurezza, in chiave proattiva, multidisciplinare e multilaterale, mediante soprattutto una maggiore convergenza di intenti a livello internazionale e il dispiegamento di strategie sinergiche ed azioni integrate di carattere diplomatico, politico, economico, di cooperazione e, in molti casi, militare. In un mondo sempre più globalizzato anche per il nostro Paese è impensabile oggi immaginare di far fronte alle minacce, anch'esse globali, limitandosi al solo presidio del territorio nazionale. Sebbene per le Forze armate resti prioritario il compito della difesa dello Stato e del territorio nazionale, di fatto, oggi la difesa e la sicurezza vengono perseguite e vengono viste anche e soprattutto attraverso la partecipazione alle varie operazioni multinazionali, di proiezione, presenza e sorveglianza nei diversi teatri operativi, nel più ampio quadro del sostegno agli sforzi della comunità internazionale, soprattutto nel contrasto al terrorismo internazionale. I fattori di crisi ed, in particolare, il terrorismo internazionale, come testimoniato in questi anni, incrementano la valenza delle operazioni internazionali per la stabilizzazione delle aree di crisi, caratterizzate da spiccata multidisciplinarietà e da connotazioni interforze e multinazionali, in cui crescente attenzione viene posta - e deve essere posta sempre più - sull'effetto sinergico del contributo militare affiancato a quelli di altra natura. il nostro Paese, nel quadro delle organizzazioni e delle alleanze di cui fa parte, fornisce un contributo importante a quel multilateralismo efficace che è e deve essere un elemento basilare della nostra azione di politica estera nell'ambito della comunità internazionale. Siamo impegnati nella gestione di aree di crisi importanti a sostegno del ruolo e del prestigio del nostro Paese e per dimostrare anche che l'Italia può costituire un valore aggiunto nell'ambito delle complesse iniziative che la comunità internazionale attua e continuerà ad attuare per la stabilità, la pace, lo sviluppo e l'affermazione ed il rispetto dei diritti umani. Rammento che l'Italia è attualmente impegnata all'estero con più di 8.000 militari, che operano in 31 missioni internazionali dislocate in 19 Paesi. Le missioni di maggiore impegno sono, nell'ordine, quelle in Afghanistan, dove operano circa 2.800 unità, nell'area dei Balcani occidentali, in cui sono impegnati più di 2.500 militari italiani, e in Libano, dove sono presenti circa 2.500 soldati. Accanto a queste sono poi in corso altre missioni che impiegano un numero minore di unità e che vedono, in alcune di esse, una partecipazione italiana che dura ed è ormai apprezzata da molti anni. Grazie alla qualità di tali contributi all'azione multilaterale, l'Italia gode oggi di un significativo prestigio nel mondo e di un apprezzamento unanime. Le caratteristiche e le dinamiche dell'attuale scenario geostrategico, pertanto, rafforzano l'esigenza per il nostro Paese di disporre di uno strumento operativo efficace, agile, integrato, proiettabile, sostenibile, a fianco e in sinergia con quelli dei principali partner internazionali, per fronteggiare le minacce esistenti, pur in presenza di una non favorevole congiuntura economica, per gestire le crisi ricorrenti, per contenere i conflitti in atto e per evitare che esplodano conflitti ancora peggiori. Si tratta di una pluralità di funzioni e di compiti che attribuiamo alla nostra politica di difesa. In primo luogo, al fine di fronteggiare le minacce esistenti, dobbiamo essere in grado di tutelare l'integrità dei nostri spazi e dei nostri interessi vitali, esercitando la nostra sovranità sul territorio nazionale, sullo spazio marittimo ed aereo, sulle vie di approvvigionamento terrestri e marittime che permettono al nostro sistema Paese di interagire col resto del mondo e della comunità internazionale. Ciò richiede la disponibilità costante di assetti militari terrestri, navali ed aerei mantenuti ad un'adeguata prontezza, idonei per numero e qualità a svolgere queste imprese in maniera qualitativamente valida. In secondo luogo, la Difesa deve essere in grado di gestire le crisi ricorrenti, siano esse di carattere politico e militare oppure di tipo umanitario, a partire da quelle che si materializzano più vicino ai nostri confini, fino alle aree metropolitane di importanza strategica. Sulla base di questo insieme di considerazioni e nella consapevolezza che vi è la necessità indifferibile di disporre di una difesa in grado di far fronte alla molteplice natura delle sfide connesse all'attuale quadro politico-strategico, è stata istituita una Commissione di alta consulenza e studio con la finalità di elaborare un disegno di legge delega per la ridefinizione complessiva del sistema di difesa e di sicurezza nazionale. Tale disegno di legge mira, tra l'altro, ad una migliore qualificazione della spesa per il comparto difesa e, di conseguenza, ad un uso efficiente delle risorse disponibili. In quest'ottica e a tal fine, è stato ritenuto utile ed opportuno fare tesoro delle esperienze e delle conoscenze che risiedono nei Dicasteri che con quello della difesa devono agire in stretta sintonia e in sinergia. È per questo motivo che tra gli attuali componenti della commissione sono stati inseriti i rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della funzione pubblica e dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ma anche dell'istruzione, università e ricerca, nonché della Presidenza del Consiglio. L'intendimento è e deve essere quello di utilizzare quale base dei lavori della commissione le indicazioni sin qui ricevute dai vertici militari e *in primis* dal Capo di Stato maggiore della Difesa, Grazie. recepisca sia le esigenze prioritarie della difesa nazionale e della partecipazione alle missioni di salvaguardia della pace e della sicurezza internazionali, sia quelle di una attenta ed efficiente utilizzazione delle risorse disponibili, cercando di ottimizzarne l'efficacia. Inoltre, così come è negli auspici degli onorevoli proponenti la mozione n. 108 (testo 2), la commissione, oltre che delle indicazioni dei vertici militari si dovrà avvalere anche di analisi, di contributi e proposte di autorità di comprovata competenza nei campi giuridico, scientifico, industriale ed economico, come pure di esperti di materie militari, della sicurezza e dell'organizzazione. Tutto ciò con l'intento e con l'obiettivo di pervenire ad una proposta di ridefinizione complessiva del Dicastero e del sistema di difesa nazionale. Ci si attende, quindi, di poter elaborare un provvedimento di legge in grado di consentire un adeguamento alle effettive esigenze attuali e del futuro, da realizzare con la necessaria gradualità, ma al contempo in tempi realisticamente brevi, e che poggi su concrete e solide basi programmatiche che vengano condivise. In tale ambito si dovrà sviluppare l'analisi e la revisione delle strutture di vertice del Dicastero in tutte le sue aree e componenti, al fine di ottenere una sempre maggiore chiarezza delle rispettive funzioni e competenze, uno snellimento delle procedure e la massima economicità di gestione. L'obiettivo primario da perseguire è quello di mantenere un ottimale livello di capacità operative dello strumento militare, in particolare garantendo qualità dei mezzi e i necessari livelli di formazione, addestramento e motivazione del personale. Occorrerà, quindi, delineare in forma più appropriata i compiti assegnati alle Forze armate, in aggiunta a quello prioritario della difesa dello Stato e a quello derivante dalla partecipazione alle missioni internazionali per la pace e la sicurezza, alla luce dei nuovi profili d'impiego delle Forze armate che si stanno ultimamente delineando, come testimoniano le recenti operazioni "Strade sicure", "Strade pulite" e l'operazione ultima, cui abbiamo assistito e che abbiamo apprezzato, per il soccorso alle popolazioni abruzzesi, denominata "Gran Sasso". Ritengo di poter concludere, sottolineando come il Governo ed il Ministro della difesa abbiano mostrato grande sensibilità verso il tema della difesa e della sicurezza, un tema di grande complessità e delicatezza per l'oggi, ma anche e soprattutto per il domani del Paese. Questo tema deve essere affrontato non senza tener conto del più ampio requisito di compatibilità con il più generale complesso e difficile quadro economico-finanziario, alla luce della non favorevole congiuntura economica. L'iniziativa del Ministro della difesa di istituire una Commissione di alta consulenza e studio è una testimonianza tangibile di questa sensibilità e di un'attenzione particolare alla tutela del bene e degli interessi dei cittadini, in quanto solo attraverso Forze armate in grado di poter fronteggiare adeguatamente le molteplici minacce che lo scenario politico-strategico

riscontriamo ogni giorno come la forte crisi economica che sta segnando questo periodo storico sia causa di recessione della quasi totalità dei settori produttivi del nostro Paese. Ma in aree del pianeta meno stabili della nostra le conseguenze della crisi si manifestano con l'inasprirsi dei disordini socio-politici, finendo con l'incrementare fenomeni quali la migrazione incontrollata, l'aumento di traffici di ogni tipo e atti di matrice terroristica. L'Italia, come sapete, è uno dei principali attori mondiali della scena politica estera e di sicurezza internazionale, trovandosi ad agire proprio in quei Paesi dove gli scontri e le violenze sono più frequenti e dove la democrazia non è ancora un diritto comune. Il nostro Paese si è sempre distinto nel settore della difesa nazionale e sul piano internazionale, ottenendo ragguardevoli risultati durante le missioni internazionali a cui ha preso parte, non senza aver pagato con pesanti perdite, anche fra i suoi stessi uomini. Premesso ciò, colleghi, la scelta dell'Italia dei Valori di presentare la mozione messa al voto oggi deriva da alcune considerazioni sui notevoli tagli apportati durante questo ultimo anno, soprattutto tramite il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tagli, colleghi, che non hanno tardato a far sentire il loro peso sull'intera macchina operativa della funzione difesa. Si sono registrate situazioni di forte criticità, che riguardano indistintamente i settori del personale, dell'esercizio e degli investimenti. I livelli di addestramento e di prontezza dello strumento militare hanno subito cali notevoli. In particolare, si riscontrano: ridotti livelli di efficienza e della disponibilità operativa di mezzi e sistemi; ridotti livelli di scorte di materiali, combustibili e dotazioni (paradossalmente siamo muniti di carri armati che non camminano, navi che non navigano e aerei che non volano per mancanza di combustibile); incremento della situazione debitoria delle spese obbligatorie; ridotte capacità operative delle Forze armate al di sotto degli standard NATO. Se l'addestramento risente di questa critica situazione, aumenta il rischio per la stessa incolumità del personale quando impegnato in teatri operativi (d'altronde, se non si fanno esercitazioni non si saprà come comportarsi durante le operazioni). L'organico dei carabinieri, inoltre, risulta sottostimato di 7.200 unità, secondo quanto riportato dal Ministro della difesa, onorevole La Russa. Che dire poi della situazione in cui versano le strutture delle Forze armate a causa della mancata manutenzione degli immobili? Alcune di esse stanno letteralmente cadendo a pezzi, anche quelle di prestigio e di immagine, oltre che quelle sede di comandi operativi. Vorrei, poi, colleghi, richiamare la vostra attenzione sul fatto che, in seguito al secondo conflitto mondiale, la maggior parte delle infrastrutture militari presenti sul territorio nazionale sono state localizzate, e sono tuttora concentrate, nelle Regioni del Centro, del Nord e, soprattutto, del Nord-Est dell'Italia. Questo fattore - sommato al fatto che, in seguito al passaggio da un esercito di leva a un esercito professionale, ad arruolarsi sono soprattutto giovani del Sud e delle Isole - comporta che la gran parte del personale militare presti servizio lontano dalle Regioni di appartenenza, con tutti i disagi che ne derivano. Negli ultimi mesi, gli organi d'informazione hanno più volte annunciato l'intenzione di chiudere e/o dismettere diverse caserme e arsenali oggi operanti, di cui buona parte situati nelle aree centro-meridionali del Paese, così che a restare danneggiato sarà ancora una volta il Sud, già penalizzato sotto tanti aspetti. Alla luce di tali presupposti, la mozione dell'Italia dei Valori impegna il Governo a procedere, con le più opportune iniziative legislative o con atti di indirizzo, verso un riassetto delle Forze armate particolarmente attento alla necessità di operare con programmi cosiddetti interforze, al fine di generare delle economie di gestione e maggiore efficienza nei settori del supporto tecnico, logistico e amministrativo, permettendo al contempo alle singole Forze armate di salvaguardare le proprie peculiarità quando eccellenti. a prevedere appositi e ulteriori finanziamenti: per permettere lo svolgimento delle missioni internazionali cui l'Italia partecipa; per dare impulso a una politica per la casa in favore del personale militare, con particolare riguardo per i centri urbani molto grandi e le città metropolitane, al fine di ridimensionare il fenomeno del pendolarismo che incide sensibilmente sulla qualità della vita dei militari e delle loro famiglie; per garantire efficaci programmi di esercitazione e aggiornamento delle professionalità e dello strumento militare; per prevedere lo studio e la programmazione di una ridislocazione delle infrastrutture militari, dal Centro-Nord al Sud del Paese, al fine di adeguare le nuove esigenze di difesa e sicurezza al nuovo contesto nazionale ed europeo, oltre che fornire garanzie di impiego dei militari presso i bacini geografici di reclutamento; per poter fare ricorso a ogni iniziativa utile a garantire e, in futuro, a implementare, la presenza di strutture e infrastrutture operanti soprattutto nel Mezzogiorno del Paese, al fine di evitare che il ridimensionamento infrastrutturale già in atto non si trasformi in un abbandono da parte dello Stato delle zone meridionali del Paese, valutando anche la possibilità che le caserme delle Forze armate oggi operanti, ma destinate all'imminente chiusura, possano essere eventualmente convertite in un supporto allo svolgimento dei compiti e degli impegni sempre più numerosi della Protezione civile.

fine degli anni Ottanta, che affidava al Parlamento ruoli davvero minoritari, di seconda e terza battuta, per ciò che riguardava tutto il problema della programmazione pluriennale dei sistemi di difesa.

ha preso avvio dall'amministrazione militare e dalle responsabilità parlamentari, ma è diventato tema di discussione di tutta la Nazione.

ed infine di affrontare contestualmente tutta la questione che attiene al fattore umano, all'Esercito come classe dirigente, alla sua formazione e al futuro possibile da noi possibile da noi pianificabile nel contesto europeo ed internazionale. Non avremo più un'altra occasione nei prossimi anni.

anch'io ho sottoscritto.

Viceversa, con quella mozione si è voluto presentare un testo che, mentre indica tra le premesse e i *considerata* molte valutazioni corrette e condivisibili, anche perché semplicemente corrispondenti ai dati obiettivi e agli elementi che in molte occasioni ci siamo scambievolmente riferiti, ha poi invece voluto inserire dati non corretti e non corrispondenti al vero. Così, ad esempio, si è voluto far riferimento ai cosiddetti tagli al bilancio della Difesa,

il periodo del recente Governo Prodi, né naturalmente di quelli precedenti, e fingendo di dimenticare che questi cosiddetti tagli sono comunque correlati ad azioni di contenimento della finanza pubblica che riguardano innanzitutto le conseguenze della nota crisi internazionale che attanaglia tutto il mondo e certamente anche i bilanci pubblici del nostro Paese. Dall'altro lato, si è voluto attribuire a questa Commissione di alta consulenza,

di ridefinizione, rimodulazione e di valutazione sull'efficienza, efficacia e attualità della presente condizione dello strumento militare nazionale. Ci si basa quindi su ipotesi; anzi, in certi casi si fa riferimento a determinati dati, dando per scontato che che vengano assunte iniziative che avranno ripercussioni sul contenimento dei costi soltanto nel medio e lungo termine; indicazioni e iniziative che non conosciamo semplicemente perché ancora non sono state

(testo 2), di cui è prima firmataria la collega Pinotti, perché ne condividiamo l'analisi e le proposte, e perché credo che partiamo tutti, Gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, dallo stesso assunto, cioè dal fatto che le Forze armate rappresentano non solo simbolicamente l'unità nazionale, ma sono, per definizione, l'espressione e l'immagine del nostro Paese un potente strumento di politica estera, a disposizione non solo del Governo, ma anche del Parlamento. Non credo di poter essere smentito nel dire che la nostra politica estera non sarebbe la stessa senza l'apporto delle Forze armate, che in questi ultimi anni, nonostante fosse in atto il loro riordino e fossero interessate da parecchi tagli, hanno dimostrato di saper rispondere con efficacia a tutte le richieste del Paese, ricevendo apprezzamenti in ambito interno ed internazionale e quindi dando corpo, sostanza ed efficacia alla politica estera dell'Italia. Esse sono strumento di pacificazione e di solidarietà internazionale e garantiscono la nostra presenza nel sistema delle alleanze internazionali e negli organismi come l'ONU, la NATO e l'Unione europea. Quando ci capita di parlare delle Forze armate - e ci succede spesso nella nostra quotidianità - lo facciamo con orgoglio, consapevoli del ruolo che i nostri militari svolgono nello scacchiere internazionale, in particolare nelle zone più martoriate, nelle aree di crisi e di rischio. I teatri che vedono protagoniste le nostre missioni sono cruciali per gli equilibri e la stabilità del mondo e dell'Italia. Per le ragioni appena citate, le Forze armate non devono essere oggetto di strumentalizzazioni, né essere tirate in questo o quel interesse di parte.

presentato in Parlamento dal Ministro, e in atti redatti dalle Commissioni esteri e difesa in occasione dell'audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa, vogliamo capire se l'impegno qualitativo e quantitativo del nostro strumento militare nazionale è così insostituibile come presidio di sicurezza ed irrinunciabile condizione per la stabilità e vorremmo capire come ciò possa conciliarsi con la politica della progressiva riduzione degli stanziamenti condotta da questo e da altri Governi. La necessità di assolvere alle esigenze di difesa, di stabilità e di sicurezza, che è conclamata nel nostro Paese, diventa cruciale e fondamentale per esso in relazione alla posizione assunta nella comunità internazionale ed in rapporto alle alleanze liberamente sottoscritte. È noto che con la fine della Guerra fredda è cambiato il modo di intendere la sicurezza su scala globale a causa dell'emergere di minacce asimmetriche come il terrorismo e del notevole impatto delle crisi internazionali su teatri lontani dall'Italia. Oggi c'è bisogno di un approccio multinazionale integrato, che risponda alle crisi non solo militari, ma anche di natura politica, diplomatica ed economica, ed è impossibile per l'Italia sottrarsi dall'esercitare un proprio ruolo nell'ambito delle organizzazioni di cui è parte. l'apparato delle Forze armate, che ha molteplici necessità, in quanto costituito da personale, strutture logistiche ed armamenti, comincia ad entrare in crisi e ciò deve preoccupare il Parlamento nazionale e deve farlo riflettere su cosa fare e su come farlo. Soprattutto quando esigenze discendenti da scenari operativi impegnano le nostre Forze armate a rispettare standard qualitativi imposti dalla normativa dell'Unione europea, dalla NATO Detti requisiti si traducono in concreti e misurabili parametri legati alla quantità e all'efficienza operativa delle risorse disponibili, ovvero del personale, delle basi, nonché dei mezzi, delle strutture e delle infrastrutture operative. Essi sono l'unica garanzia di interoperabilità, di efficacia e di diminuzione del rischio di perdita di vite umane. Il bilancio della Difesa è quindi lo strumento in cui la volontà politica e le capacità militari devono trovare una realizzazione compiuta, in coerenza con gli impegni operativi richiesti sia sul territorio nazionale che all'estero. La legge n. 331 del 2000, che ha introdotto il modello cosiddetto professionale, prevedeva un'entità complessiva di 190.000 unità per Esercito, Marina ed Aeronautica e una loro ristrutturazione e riorganizzazione anche territoriale.

e del 40 per cento nel 2010, con evidenti ripercussioni sulla effettiva realizzabilità di quanto a suo tempo deciso in Parlamento. La conseguenza è una progressiva riduzione nel 2009 dei reclutamenti, destinati a diventare pressoché nulli dal 2010, in attesa dell'avvenuto esodo del personale più anziano. Questo implicherebbe una sospensione per anni del sistema scolastico delle Forze armate ed un invecchiamento dello strumento militare. Si tagliano anche le spese di esercizio, che, per chi non lo sapesse, finanziano l'addestramento: meno esercitazioni per l'Esercito, meno ore di navigazione per la Marina, meno ore di volo per l'Aeronautica; impossibilità di assolvere a tutti i compiti operativi e, soprattutto, diminuzione dei margini di sicurezza nell'impiego, giacché minore l'addestramento maggiori sono i rischi. La conseguenza di tutto ciò è che le Forze armate diventano più vecchie e meno addestrate. Non solo, ma si tagliano anche gli investimenti, ovvero il rinnovamento di mezzi e materiali, l'ammodernamento e 1'adeguamento tecnologico degli armamenti, indispensabili in condizioni di operatività sempre più difficili. Mi riferisco, ovviamente, alle missioni internazionali. Con una sola parola, quindi, si diminuisce anche la sicurezza del personale militare impegnato nelle missioni all'estero e sul territorio nazionale.

Sorge, allora, una domanda: se vengono introdotti questi tagli così consistenti, cosa si pensa di fare delle nostre Forze armate? Non è pervenuta infatti al Parlamento una modifica della legge n. 331 del 2000 e, quindi, si accetta, da un lato, la consistenza organica ed il modello organizzativo da essa proposti e, dall'altro, un decadimento delle attuali capacità operative e dell'efficienza delle Forze armate, che ciò sia accompagnato da una nuova riflessione, anche in ragione delle ridotte disponibilità economiche, sulla validità del modello a suo tempo approvato e sul ruolo che l'Italia vorrà assumere nei prossimi anni nel contesto internazionale. Non è accettabile che attraverso provvedimenti di natura prettamente finanziaria - e questo è il cuore politico della mozione proposta dai colleghi del PD, che sosteniamo si modifichi l'assetto della Difesa a suo tempo varato dal Parlamento. È necessario accompagnare la riduzione degli stanziamenti, se si intende continuare su questa strada, con una riorganizzazione del modello di difesa, altrimenti la situazione è dettata solo ed esclusivamente dall'inerzia. Non siamo, per la verità, da soli a denunciare questo stato di decadimento della struttura militare; anche il Ministro della difesa nel documento di accompagnamento al bilancio ha usato parole molto forti. Egli ha, infatti, affermato che, nell'ambito del settore del personale, i vincoli posti dal decreto-legge n. 112 del 2008, che stabilisce - come si è detto - una riduzione del 7 nel 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010 delle risorse a suo tempo destinate alla professionalizzazione, modificano sostanzialmente i parametri del modello professionale. Infatti, a fronte delle 190.000 unità di personale per le tre Forze armate si potrebbe arrivare, in assenza di interventi correttivi sul 2012 (anno di entrata a pieno regime del decreto-legge n. 112), ad una consistenza complessiva di 141.000 unità. Portare repentinamente le Forze armate a 140.000 unità, con un letterale sconvolgimento del modello recentemente approvato, significa far saltare tutti gli accordi internazionali che il nostro Paese ha liberamente concluso, per non parlare degli accordi bilaterali che l'Italia sottoscrive in chiave di cooperazione e di assistenza con tanti Paesi. Si pensi al Kosovo, al Corno d'Africa e a tante altre realtà in cui siamo protagonisti nello scenario internazionale. Mi chiedo se l'Italia sarebbe disposta a fare ciò, ovvero a rivedere e ridimensionare il proprio ruolo nello scenario internazionale o se, viceversa, non opterebbe per confermare tale ruolo, assicurando alle Forze armate risorse e mezzi finanziari adeguati.

pur consapevoli che certe razionalizzazioni si debbano compiere colpendo sprechi, duplicazioni di funzioni e ruoli, vi è la necessità di uno sforzo comune per garantire al nostro Paese la continuità della sua azione a livello internazionale tutelando ciò che le Forze armate fino ad oggi hanno garantito: stabilità, sicurezza e pace. e pace. Una politica dei tagli che non è collegata ad una riorganizzazione del sistema in ragione delle esigenze internazionali del nostro Paese ci porta dritti a non affrontare un tema che comunque è cruciale e che questo Parlamento, anche a prescindere dalla volontà del Governo, è tenuto a fare: il Parlamento infatti, prima del Governo, ha il compito di tutelare le Forze armate come bene supremo del nostro Paese, come tutori di un interesse generale che prescinde dalle forze politiche che oggi governano e quelle che oggi stanno all'opposizione.

ogni qual volta si parli di difesa o di necessità di affrontare tutto ciò che attiene alla difesa, cioè una riforma radicale. Tale riforma deve deve tenere in considerazione, almeno per quanto riguarda storicamente i radicali, due dimensioni: la necessità di promuovere una difesa europea nonché una progressiva

Voglio citare, signora Presidente - la ringrazio, anzi, per averli più volte fatti emergere in dibattiti pubblici - dei dati elaborati da un pensatoio, che ha sede nel Regno Unito e che si chiama *The European Council on Foreign Relations,* relativamente a tutto ciò che attiene ad una comparazione tra difesa europea e difesa statunitense. La spesa militare degli Stati membri dell'Unione europea ammonta a 201 miliardi di euro, di cui il è a carico di Gran Bretagna e Francia. Complessivamente il 55 per cento di questo bilancio serve per mantenere quasi 2 milioni di uomini e donne in uniforme. Gli USA spendono solo il 20 per cento del proprio bilancio militare per spese di personale; viceversa, spendono il 29 per cento del proprio bilancio per investimenti, approvvigionamento di armi, ricerca e sviluppo, mentre gli europei vi dedicano solo il 19 Più significativo ancora è il fatto che solo il 30 per cento del personale europeo è in grado di essere dispiegato all'estero: resta un mistero che cosa faccia il rimanente 70 per cento. Ma la percentuale mobilitabile, già di per sé bassa, diventa ancor più piccola, perché, di fatto, non viene neanche questa tutta dispiegata: nel 2006, solo 98.000 unità, cioè circa il 5 per cento del totale, sono state inviate all'estero, incluse operazioni che non hanno a che fare con la PESD, in Afghanistan e Libano.

e della stabilità internazionale quanto più possibile sotto l'egida delle Organizzazioni regionali o internazionali, come l'Unione europea stessa ma anche le Nazioni Unite; partecipazione

non propriamente positiva: la nostra partecipazione alla produzione di 131 cacciabombardieri F-35, che ci costeranno 15 miliardi di euro.

anche perché in esse si sostiene un'esigenza primaria, importante, come la difesa nazionale.

Oggi, per lo più, difesa nazionale vuol dire essere presenti in missioni all'estero, chiamate missioni di pace, missioni di stabilizzazione. Infatti, l'Italia è presente in 19 Paesi negli scenari più diversificati,

difesa nazionale contrapposta al rischio di aggressione non sia più quella tradizionale. Ormai il nemico non si affronta più *de visu,* perché il nemico non ha più un viso; il nemico è ormai invisibile. Il nemico per tutti i Paesi occidentali è il terrorismo internazionale,

I tagli lineari hanno probabilmente risolto un problema di emergenza finanziaria che rispondeva ad esigenze di carattere generale.

o, magari, anche all'interno dello stesso Dicastero, le varie strutture responsabili avrebbero preferito che altre facessero sacrifici

Signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli senatori, la discussione sulle Forze armate è un'occasione preziosa perché raramente aspetti importanti concernenti la difesa sono oggetto di approfondimento in quest'Aula. Anche l'impiego nelle operazioni internazionali, che come sappiamo perfettamente rappresenta l'espressione forse più evidente della nostra politica estera, è sottoposto solo parzialmente alle valutazioni di quest'Assemblea. Il Parlamento esamina essenzialmente gli aspetti finanziari senza dar vita ad un ampio e credo doveroso confronto sulle singole missioni. quindi a mancare quella discussione che consentirebbe di esprimere indirizzi politici sulle operazioni, di valutare i risultati conseguiti e di approfondire gli aspetti relativi alle missioni più delicate. In questo quadro di limitato coinvolgimento del Parlamento sugli aspetti rilevanti della Difesa, la mozione n. 108 (testo 2) sulle Forze armate acquista notevole importanza. Ci consente infatti di ricordare le criticità dello strumento militare: un organismo che richiede pianificazioni a lungo termine e che ha bisogno di risorse adeguate e costanti nel tempo. Queste ultime sono parole del Ministro della difesa, nel giugno 1995, che purtroppo, e direi clamorosamente, sono state successivamente disattese dai successivi atti del Governo. un organismo che non è in grado di sostenere drastiche riduzioni di risorse che non siano collegate a proporzionali diminuzioni dei compiti da assolvere. La percentuale dello 0,85 del prodotto interno lordo, assegnata al comparto della Difesa per il 2009, contrasta in maniera stridente con le parole dell'allora Ministro della difesa e, nella graduatoria dei fondi per le Forze armate, colloca l'Italia nel gradino più basso tra i Paesi con i quali normalmente cooperiamo e ci confrontiamo. I tagli al bilancio della Difesa hanno effetti negativi su tutto il settore e ciò non può non preoccuparci. Per quanto attiene all'esercizio, quei tagli limitano le possibilità di intervento e di manutenzione delle infrastrutture, abbassando le condizioni di vita del personale; influiscono pesantemente sulla disponibilità delle scorte; soprattutto, incidono, in misura fortemente riduttiva, sulla preparazione del personale e delle unità, si contrae il numero delle esercitazioni, quello delle ore di volo e delle attività in mare. In definitiva, diviene difficile mantenere i livelli di efficienza operativa e le capacità logistiche indispensabili. rischia di essere posta in discussione la stessa strategia seguita negli ultimi anni dal Paese di partecipazione alle più importanti missioni internazionali e di sostegno all'integrazione europea. Altrettanto penalizzanti sono le riduzioni delle risorse destinate al settore del personale. La consistente entità dei tagli operati (il 7 per cento nel corrente anno e il 40 per cento nel 2010-2011) comporterà certamente una forte contrazione degli arruolamenti dei nuovi volontari e un'insufficiente immissione di giovani in un organismo sempre più composto da persone anziane. Ne risulterà pesantemente condizionato tutto il processo di professionalizzazione e, all'interno della struttura, il bilanciamento tra le varie categorie. Le preoccupazioni di cui sto parlando non possono essere sottovalutate sono le stesse preoccupazioni di tutti i massimi responsabili della Difesa a livello tecnico, del Capo di Stato maggiore della Difesa e dei Capi di Stato maggiore delle diverse Forze armate, che in più circostanze hanno paventato una diminuzione dell'efficacia e delle capacità operative dello strumento. Si tratta di preoccupazioni che rendono ancora più incomprensibile l'atteggiamento dell'Esecutivo, che da una parte opera tagli di entità mai raggiunta in precedenza alle risorse finanziarie destinate al comparto difesa, e dall'altra impegna aliquote sempre più consistenti delle Forze armate in compiti non prioritariamente di loro competenza. Sono preoccupazioni, infine, che attengono anche al possibile ridimensionamento della struttura militare: da più parti è stata avanzata l'ipotesi che la Commissione di alta consulenza, di cui abbiamo già parlato, per l'esame della problematica (di cui peraltro finora non conosciamo gli aspetti), possa giudicare, sulla base delle risorse destinate alla Difesa, non più sostenibile il modello a 190.000 unità. Vorrei ricordare che il suddetto modello, stabilito da una legge del Parlamento (la legge n. 331 del 2000), derivava da chiari indirizzi politici in merito al livello di presenza dell'Italia nel contesto internazionale da ben definite prospettive di partecipazione agli impegni delle alleanze e alle operazioni di stabilizzazione delle aree di crisi. Era, in sostanza, un modello di difesa perfettamente giustificato in ogni sua parte ed armonico nel suo complesso. Per questi motivi, la mozione a prima firma Pinotti si prefigge innanzi tutto lo scopo di impegnare il Governo in merito alla necessità di salvaguardare l'efficienza delle Forze armate, garantendo il flusso di risorse finanziarie adeguate, ma vuole anche evidenziare l'esigenza del coinvolgimento del Parlamento nell'eventuale modifica del modello a suo tempo approvato dalle Camere. Per quanto riguarda il primo aspetto,

quali chiedevano e chiedono al Governo di ripristinare le assegnazioni necessarie per il 2009 e di annullare le riduzioni già decise per gli anni futuri. Ciò purtroppo non è ancora avvenuto e le Forze armate continuano a subire questa penalizzante situazione. In merito al secondo aspetto, ossia la possibile razionalizzazione della struttura, qualora emerga la volontà di rivedere il modello a 190.000 unità, nessun provvedimento risulterà appropriato, se non saranno stabiliti preventivamente determinanti aspetti di politica militare. Bisognerà decidere - com'è avvenuto nell'anno 2000 per il modello di difesa attualmente in vigore - quale livello di presenza l'Italia voglia esercitare nel contesto internazionale; valutare se deve proseguire l'integrazione delle sue Forze armate nel contesto dell'Europa, così com'è avvenuto finora; decidere se partecipare alle operazioni di supporto alla pace, com'è stato fatto fino ad oggi; definire infine i principi per la riconfigurazione del nuovo strumento sulla base delle caratteristiche dei possibili impegni operativi. Credo che il Parlamento non potrà non essere pienamente coinvolto in queste decisioni; il Partito Democratico è disponibile è disponibile a valutare tutti gli elementi di possibile recupero delle risorse e di risparmio di spesa, ricordando naturalmente che le Forze armate sono una parte importante del nostro Stato e che il personale che opera, vive e e lavora all'interno di questa struttura deve essere valorizzato e non mortificato. Signora Presidente, onorevoli colleghi, questo dibattito su mozioni d'indirizzo a favore del settore della Difesa si svolge alla vigila del G8 dell'Aquila; un appuntamento importantissimo per le decisioni che dovranno essere assunte e nel quale il nostro Paese metterà alla prova quel prestigio di cui oggi gode meritatamente nel mondo e che le Forze armate hanno contribuito ad affermare, fornendo un serio ausilio, in termini di efficienza e professionalità, a quel multilateralismo efficace che è elemento basilare alla nostra azione di politica estera nell'ambito della comunità internazionale. Questo dibattito, però, precede anche l'invio in Afghanistan della prima parte di quel contingente di 500 unità aggiuntive che il Governo italiano ha deciso di schierare a protezione del processo di pace nel delicato frangente delle elezioni presidenziale di quel Paese. Una scelta coraggiosa, presa con grande senso di responsabilità, che onora la nostra collaborazione con la NATO e l'ONU e che riconferma concretamente la nostra vicinanza agli alleati statunitensi impegnati in questi giorni in duri combattimenti contro formazioni qaediste e talebane nella provincia meridionale della valle dell'Helmand. Ecco perché, cari colleghi, ritengo che, nell'odierna discussione, dovremmo riuscire a far prevalere le ragioni dell'interesse e della solidarietà nazionale sulle facili, ma sterili, polemiche di parte (per altro - intendiamoci - legittime, anche quando strumentali). Lo dico in particolare ai colleghi dell'opposizione, il cui apporto critico e propositivo in Commissione difesa ho sempre apprezzato. Vedete, colleghi, se una critica ai tagli operati dal Governo vuole esprimere preoccupazione per la tenuta della capacità operativa delle Forze armate, servendo così da stimolo per giungere ad assicurare, tutti insieme e nel tempo, stabilità e coerenza all'assegnazione delle risorse necessarie al comparto della Difesa, essa può essere tranquillamente compresa. Se tale critica invece vuole sottintendere un disinteresse del Governo, magari accompagnato dalla volontà di penalizzare le Forze armate, allora non può che essere respinta con la massima fermezza, perché ignora volutamente un dato di sistema, e cioè che tagli a spese e investimenti sono stati effettuati in tutti i settori della pubblica amministrazione, in conseguenza delle restrizioni imposte al bilancio dello Stato, non da una qualsiasi congiuntura, ma da una terribile crisi economica di natura globale e di carattere epocale, e perché ignora volutamente un dato storico, quello della vicinanza etica, culturale e ideologica del centrodestra alle Forze armate, che difendevamo, colleghi del centro-sinistra, quando altri le insultavano, bruciandone talvolta i simboli o aggredendone gli uomini in uniforme, come è avvenuto nel nostro Paese in un passato ancora troppo recente. Una vicinanza, la nostra, che si fonda - storicamente - sui valori patriottici, valori difesi dalla schiacciante maggioranza dei cittadini con il loro lavoro, e quelli difesi dalle stesse Forze armate, la cui evoluzione (da esercito di popolo a esercito di professionisti) il Governo Berlusconi, o meglio, i Governi Berlusconi hanno saputo favorire e sostenere sempre in un ruolo di pace in Italia e all'estero, nell'interesse della Nazione italiana e nel quadro del suo sistema di alleanze. Vorrei che vi fosse più considerazione per gli sforzi compiuti nel realizzare, senza alcun danno sociale, il passaggio dalla leva obbligatoria al professionismo militare; così come, naturalmente, vorrei vi fosse più considerazione per i problemi che tale trasformazione ha posto e pone: in termini di costi e gestione del personale, di aggiornamento e razionalizzazione dei modelli organizzativi e di costruzione di un efficace rapporto, fra investimenti diretti alla Difesa e lavoro per l'indotto industriale della Difesa, nell'ambito di un quadro di programmazione e compatibilità economica. Sono tutte problematiche che verranno comunque affrontate dalla Commissione di alta consulenza istituita dal ministro La Russa, Commissione che dovrà informare tempestivamente il Parlamento prima dell'avvio dell'*iter* di approvazione del disegno di legge delega per la ridefinizione complessiva del sistema di difesa e sicurezza nazionale; in modo che la ricerca del massimo di condivisione possibile possa accompagnare la ferma assunzione di responsabilità politica che compete a chi deve prendere decisioni atte a riformare il sistema di difesa italiano, sull'esempio di altri Paesi europei nostri alleati nella NATO. Vorrei però ritornare sulla polemica relativa ai tagli per alcune doverose precisazioni e per insistere sul rapporto tra politica della difesa e politica dell'economia, ai fini della sicurezza nazionale ed internazionale. È bene precisare, intanto, proprio a partire dai profili di interesse per il comparto Difesa presenti nel bilancio 2009 dello Stato, che l'inevitabile contrazione degli stanziamenti su alcuni capitoli di spesa - sottolineata 108 (testo 2), Pinotti ed altri - risulta sostanzialmente compensata da importanti impegni formalmente afferenti ad altri Ministeri eppure direttamente connessi alle esigenze delle Forze armate. Ricordo lo stanziamento, da parte del Ministero dell'economia, di un miliardo di euro relativo al Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace. Ricordo i 565 milioni di euro destinati al Fondo per le spese riservate ai servizi di informazioni e di sicurezza sia civili che militari; i 380 milioni di euro erogati dal Ministero dello sviluppo economico per il Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese da destinarsi all'industria aerospaziale; il miliardo e 360 milioni di euro destinati a interventi agevolativi per il settore aeronautico, ai quali vanno aggiunti i 180 milioni per l'acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione), ricompresi poi nel Programma di incentivazione per lo sviluppo industriale. Senza dimenticare che, all'interno del disegno di legge recante delega al Governo in materia di lavori usuranti, è prevista una norma di notevole interesse per la Difesa, relativa - cito testualmente - «al riconoscimento di specificità delle Forze armate ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica pensionistica e previdenziale». L'importante è non considerare la politica dell'economia con i provvedimenti di rigore gestionale, che essa può imporre al fine di ricreare le condizioni di uno sviluppo, come ostativa al potenziamento dei sistemi di difesa. Perché, da sempre, i due requisiti essenziali di una società in evoluzione sono una consolidata base materiale e un'adeguata sicurezza. E, da sempre, l'arte strategica punta a dare sicurezza alla società, senza pregiudicare la vitalità delle sue basi economiche. Concludo allora con una citazione di McNamara, il grande Segretario alla Difesa degli Stati Uniti scomparso proprio ieri. diceva: «Nel mondo moderno la difesa nazionale, la sicurezza saranno rappresentate sostanzialmente dallo sviluppo economico e scientifico. Talvolta è difficile comprenderlo, per noi che abbiamo vedute un po' stereotipate, che calcolano la sicurezza in termini puramente militari. È chiaro che la sicurezza ha aspetti militari ma commetteremmo un errore pericoloso considerando anche in futuro come sinonimi potenza militare e sicurezza. Una delle maggiori follie nella storia dell'uomo è costituita sempre nello spendere di più per procurarsi i mezzi per fare le guerre, che per assicurarsi quelli capaci di evitarle». Grazie.

caso, il signor Sottosegretario o, comunque, intervenendo nel dibattito, abbiano voluto significare l'importanza che si vuole dare al comparto della difesa in questo momento particolare. Il senatore Gamba ha parlato anche di un'occasione perduta. Da questo punto di vista il Governo non può che rammaricarsi del fatto che, pur in presenza di moltissime sovrapposizioni di una visione sostanzialmente condivisa su aspetti molto importanti presenti in tutte le mozioni per una serie di motivazioni legittime e che naturalmente differenziano le singole forze politiche, non si sia pervenuti ad un unico che avrebbe avuto maggiore forza nel suo essere condiviso. Da questo punto di vista, penso sia opportuno che il Governo esprima il proprio parere su ogni singola mozione

l'azione del Governo debba essere valutata nella sua pluralità. Le forze politiche si sono assunte la responsabilità di indicare, anche attraverso le premesse e i *considerata*, la

Pinotti, che contiene in larga parte, e nelle premesse e negli impegni, una visione che il Governo ritiene essere propria, tuttavia non è condivisibile nel suo insieme e in particolare non

in maniera ovviamente semplificata, ma non semplicistica, "tagli" apportati al bilancio della Difesa. non disconosce il suo intento di riforma e intravede quelli che possono essere definiti tagli e che tali appaiono in una visione semplificata,

dei cardini dell'attività di Governo. Si vuole cioè ottenere un maggiore efficientamento della spesa pubblica attraverso un maggiore efficientamento dell'azione di ogni amministrazione pubblica. Questo vale per tutte le amministrazioni e anche per Di conseguenza, quando si parla semplicemente di tagli, ebbene, noi riteniamo non si voglia rendere merito ad un'azione del Governo di ben più ampia portata. Voglio far riferimento ad alcune questioni, peraltro esplicitate anche nel corso degli interventi. È stato affermato che il disposto del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133, avrebbe previsto per l'arruolamento un taglio del 40 a partire dal 2010. Più correttamente, come peraltro recita la norma, il taglio previsto, di cui il Governo non ha difficoltà a riconoscere l'utilità ai fini dell'efficientamento, è del 7 Il restante 33 per cento è da ottenersi attraverso una riduzione di costi all'interno del bilancio. se l'amministrazione non fosse in grado di ottenere altri risparmi, il disposto agirebbe sull'arruolamento; ma dire che il taglio è del 40 per cento equivale a sostenere che l'amministrazione della difesa, in particolare le Forze armate, non saranno in grado, attraverso un efficientamento della loro attività, di produrre i risultati che il Governo si è prefisso.

è il principale sottoposto e consigliere del Ministro della difesa, ha parlato di un pericolo ovvero di un rischio, non ha parlato di quello che accadrà bensì di ciò che accadrebbe se il combinato disposto dell'azione politica del Ministro e dell'azione amministrativa delle Forze armate rendesse impossibile il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento che ci siamo posti. Dire che il Capo di Stato maggiore ha descritto le Forze armate del futuro è dire che il Capo di Stato maggiore e le Forze armate non saranno in condizione di avvicinarsi neanche agli obiettivi di efficientamento che il Governo ha realizzato, e questo per il Governo non è tollerabile. Il Capo di Stato maggiore della Difesa e le Forze armate stanno lavorando con grande attenzione per fare la loro parte - e siamo un'amministrazione virtuosa - nell'ottica dell'efficientamento e della riduzione della spesa. Non è accettabile neanche la visione che viene data del cosiddetto modello a 190.000 uomini. Quando si dice che che toccando quel modello si stravolge il sistema difesa del nostro Paese, si fa torto alla realtà. Come tutti sanno - e come il senatore Del Vecchio sa meglio di altri - quello è un modello teorico che prevedeva un'evoluzione nel tempo nel corso di 15 o 20 anni. Non ho difficoltà ad affermare in quest'Aula che le Forze armate italiane, dopo l'approvazione della legge n. 331 del 2000, non hanno mai raggiunto i 190.000 i 190.000 uomini. La forza bilanciata, ovvero il numero di soldati realmente presenti, è sempre stata inferiore. Non ho difficoltà a confermare in quest'Aula che, poiché il modello a 190.000 uomini partiva da una situazione di professionisti che doveva reggere un esercito di 300.000 uomini, inizialmente prevedeva un numero di quadri non più impiegabili per attività operative nell'ordine delle 30.000 unità;

superiore nel totale ai 12.000 uomini - ha sempre fatto riferimento a un totale per le tre Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di militari impiegabili in attività operativa mai superiore ai 150.000 uomini. Ciò significa che questo Governo e quelli che lo hanno preceduto sono riusciti a garantire la partecipazione italiana a missioni internazionali per un livello medio superiore ai 12.000 uomini, con una disponibilità operativa inferiore ai 160.000 uomini. Non citiamo come un feticcio 190.000 uomini; parliamo di obiettivi, di capacità, di volontà politica. non è accoglibile anche nella visione che vuole proporre della, più volte citata in quest'Aula, Commissione di alta consulenza e studio per la ridefinizione complessiva del sistema di difesa e sicurezza

il Ministro della difesa ha comunicato che, come primo passo interno della sua amministrazione verso la futura riforma globale del sistema di Difesa, che include anche la riorganizzazione delle Forze armate e del suo Ministero,

Grazie, Presidente. Dire poi che il Parlamento e i parlamentari non sanno abbastanza dell'attività della commissione pare essere in parziale contrapposizione con il fatto che alla commissione vengono attribuiti ruoli insufficienti e mancanze nella composizione. Il Parlamento correttamente non conosce ancora quello che questa commissione sta facendo: criticarla senza sapere come sia organizzata mi sembra un atteggiamento politicamente rispettabile, ma che il Governo non può accettare. Da questo punto di vista, la ragione per cui ancora il Parlamento non sa niente di questa commissione è insita nel fatto che si tratta di una commissione propria del Ministro della difesa, che svolge un'opera

della difesa sembrerebbe andare oltre le sue prerogative e tentare di mettere il Governo davanti al fatto compiuto di un testo di legge concordato con il Parlamento prima di aver percepito - questo sì che il Ministro della difesa lo sta facendo - la posizione delle diverse amministrazioni. È infatti evidente che il tema della Difesa non è del del Ministero della difesa, ma coinvolge il Governo nella sua interezza, dalla Presidenza del Consiglio al Ministero degli affari esteri al Ministero dello sviluppo economico, ma anche alle realtà locali. Questa è la ragione per cui ad oggi il Parlamento non ha saputo nulla. Esiste l'impegno formale da parte del Ministro, terminati i lavori della commissione e verificata la loro compatibilità con la proposta fatta in sede di Governo, di tenere informato il Parlamento ancor prima di provvedimenti che potranno avere natura legislativa, ma anche regolamentare, ovvero senza la necessità di un intervento del Parlamento. Questo sì è un impegno politico che il ministro La Russa ha preso più volte in Commissione e, in particolare, qui al Senato. nel rispetto del ruolo del Parlamento riteniamo che non possa essere fatto prima, ma comprendo che, al di là delle parole usate, questo era l'intento delle mozioni così come sono state presentate. Sono queste quindi le ragioni che riguardano sia le premesse, sia le considerazioni e, in alcuni casi, anche gli impegni - per le quali il Governo non può accogliere nella sua interezza la mozione n.

la gran parte degli arruolamenti all'interno delle Forze armate provenga dal Mezzogiorno, il che rappresenta un fatto noto. Da questo punto di vista, non sono dunque accoglibili nella loro interezza gli impegni così come presentati, perché la tempistica e le necessità della difesa

di questa amministrazione, nonché nella lettura corretta dell'iniziativa che il Ministro della difesa ha intrapreso in relazione alla Commissione di alta consulenza. Per quanto riguarda gli impegni, sono tutti condivisi dal Governo. In particolare il Governo non ha difficoltà ad accettare la possibilità di estendere il coinvolgimento di esperti di varia natura all'interno della Commissione, anche per venire incontro ad alcune tematiche - come peraltro sottolineato anche dal senatore Caforio - che legano le Forze armate alle realtà Questo problema esiste tanto al Nord quanto al Sud, che produce la gran parte degli arruolati: il Ministero della difesa quindi ben volentieri si confronterà con le realtà locali per prendere in considerazione anche questa tematica.

ho parlato di tagli, ma di proposte di efficientamento. È vero che a volte tali proposte non hanno avuto altro mezzo di esplicitarsi che attraverso tagli lineari, ma è evidente che poiché il risultato che si persegue è il reale efficientamento, differenze tra singole amministrazioni nella struttura dei costi e della spesa dovranno essere prese in considerazione, eventualmente anche in norme di carattere primario. Ciò che conta per la Difesa è che le risorse siano stabili e congrue; noi noi non ci tireremo indietro se ci verrà chiesto di efficientare la nostra attività.

così come chiaramente premesso nella mozione del Gruppo Italia dei Valori e in quella a prima firma della collega Pinotti, si sottolinea come, fin dal secondo dopoguerra, l'Italia partecipa a importanti missioni a carattere multinazionale che portano le sue Forze armate a prestare servizio fuori dai confini del Paese. Non vi è, quindi, alcun dubbio che le Forze armate italiane rappresentino un elemento indispensabile per consentire all'Italia di assumere i propri impegni impegni nell'ambito di tali organizzazioni internazionali e per portarli avanti con coerenza e successo. La responsabilità primaria della nostra politica estera e di difesa è oramai rivolta alla prevenzione, al controllo e alla stabilizzazione delle crisi che, in più zone del mondo, attentano alla pace e alla sicurezza internazionale. Purtroppo, se oggi siamo qui a votare delle mozioni sulla necessità di garantire risorse al comparto difesa è perché si rilevano già le conseguenze dovute ai tagli subiti dal bilancio della Difesa nel triennio 2004-2006 e poi aggravati da quelli previsti per il triennio 2009-2011. Occorre prendere coscienza che ad essere compromesso è il livello degli impegni e obiettivi previsti per le nostre Forze armate: saranno messi in discussione l'esercizio e i settori dell'addestramento, provocando un calo della capacità operativa delle Forze si continuerà a registrare, come già riscontrato, un calo dei livelli di efficienza e disponibilità operativa di mezzi e sistemi, e dei livelli di scorte di materiali, combustibili e dotazioni. Ad aumentare sarà solo il debito delle spese obbligatorie del settore. È quindi, assolutamente necessario che il Governo provveda a generare economie di gestione e maggiore efficienza nei settori del supporto tecnico, logistico, amministrativo, per mezzo di opportune iniziative legislative o con atti di indirizzo. Si richiedono inoltre appositi e ulteriori finanziamenti per lo svolgimento delle missioni internazionali a cui l'Italia partecipa, per garantire efficaci programmi di esercitazione e aggiornamento delle professionalità e dello strumento militare. Inoltre, non vanno trascurate voci di spesa quali quelle per gli interventi di manutenzione alle infrastrutture, ormai praticamente fermi alla prima metà del corrente decennio, e le spese utili a garantire la presenza di strutture e infrastrutture che operino nel Mezzogiorno. Laddove, poi, si dovesse procedere con la dismissione di caserme e arsenali, riteniamo opportuno considerare di destinare tali strutture all'utilizzo da parte della Protezione civile. Naturalmente, l'esteso fenomeno del pendolarismo del personale militare incide sensibilmente sulla qualità della vita degli interessati, ma anche delle loro famiglie. Ulteriori finanziamenti sono, quindi, necessari anche per lanciare una politica per la casa in favore di tale personale militare. Parimenti, nella mozione dell'Italia dei Valori è contemplato l'avvio di un progetto che si occupi della ridislocazione delle infrastrutture militari dal Centro-Nord del Paese al Sud, affinché i militari abbiano la possibilità di prestare servizio presso i bacini geografici di reclutamento.

perché riteniamo giusto cominciare a discutere di questi temi, ma non dobbiamo dimenticare che in passato le Camere non hanno avuto l'attenzione che serviva

noi non crediamo, come Partito Democratico, che quella odierna sia un'occasione perduta; anche noi, alla stessa stregua di quanto ha dichiarato il sottosegretario Cossiga, siamo del parere che vi fosse un grande bisogno di addivenire ad un'occasione, ad una opportunità dalla quale potesse discendere chiarezza,

Il Partito Democratico e l'Italia dei Valori non si sono inventati a caso la formulazione di una mozione: lo hanno fatto con estremo senso di responsabilità e, se posso dirlo, con sobrietà politica, nella speranza di ricollocare al centro il Parlamento. Signora Presidente, cari colleghi, stasera non se ne è parlato e voglio farlo io. Voglio ricordare a chi non ne avesse ancora mantenuto memoria che questa volta non ci sarà un decreto specifico sulle missioni internazionali; questa volta il Governo ha ritenuto di dover di dover immettere in un decreto *omnibus* questo argomento così importante, di fatto togliendogli quella connotazione e quella caratteristica che un argomento così importante mantiene. Come si fa da parte soprattutto del Governo, a sostenere che c'è il massimo di attenzione nei confronti del Parlamento, se in quello che può essere considerato l'unico passaggio

Sono molte le ragioni per le quali noi abbiamo timore che nei confronti di questo ambito così importante della pubblica amministrazione il Governo stia sbagliando. Siamo quelli dell'articolo 11: siamo quelli che hanno bene presente le determinazioni contenute nella Costituzione, ma siamo anche quelli che ritengono di dover tutelare e difendere l'intera pubblica amministrazione. Ed il comparto difesa e sicurezza è un pezzo prezioso della pubblica amministrazione. È stato ricordato da parte del Sottosegretario il passaggio del Capo di Stato maggiore della Difesa che, a mio giudizio, non ha bisogno di essere interpretato dal Governo. Il Capo di Stato maggiore della Difesa dice ciò che pensa. Afferma ciò in cui crede. Quest'uomo, questa alta carica dello Stato non solo ha lamentato

e paventato l'eventualità che ci si possa, come Paese, rifiutare di garantire il cambio delle missioni internazionali qualora dovessero pervenire richieste al nostro Stato che non siano ancora inserite nell'elenco in vigenza. Ecco, questa è concretezza delle cose. Nella mozione presentata dalla collega Pinotti non vi è una Noi non vogliamo accentuare l'aspetto degli scontri, ma anzi approfittiamo di questa occasione per ricordare al Governo anche a parte della maggioranza, ma fondamentalmente al Governo - che i nostri uomini, nei teatri di crisi, compreso l'Afghanistan, sono lì per essere portatori di pace. Approfittiamo dell'occasione per sottolineare che ci sembra sempre più ineluttabile, ancorché non accolta da parte nostra, una identificazione fra il programma ISAF ed il programma *Enduring Freedom*. Non possiamo accettare di essere assorbiti dal programma *Enduring Freedom* perché le regole stabilite dal Parlamento sono ferree, chiare e non possono essere bypassate per volontà di alcun tipo di Ministro. E poi trovo singolare, signora Presidente e colleghi, che il Consiglio supremo, che contiene nella propria definizione la sua importanza, nomini una Commissione di alta consulenza

il Paese, a partire dal Parlamento, potesse partecipare alla determinazione del nuovo modello di difesa. I numeri indicati dalla collega Pinotti, dai colleghi dell'Italia dei Valori e dell'UDC sono veri, non sono un'interpretazione. Desideriamo che si faccia chiarezza sul modello di difesa, che ci si dica se abbiamo ancora un modello basato su 190.000 unità oppure su 141.000, che ci vengano date garanzie sulle spese di esercizio, non perché siamo guerrafondai perché siamo ligi al dettato costituzionale e siamo più sensibili alla necessità di garantire la sicurezza dei soldati piuttosto che ad abbandonarci a forme di sentimentalismo un po' spurio

al Gruppo dell'UDC per le dichiarazioni rese dal senatore D'Alia e chiariamo che riteniamo appena aperto il discorso, perché questa, per il Partito Democratico, non è un'occasione perduta.

Signora Presidente, signor Sottosegretario, care colleghe, colleghi, il Gruppo del Popolo della Libertà voterà a favore della mozione che ho presentato insieme ai colleghi Gasparri, Bricolo, Quagliariello ed a tutti i componenti del nostro Gruppo che appartengono alla Commissione che mi onoro di presiedere. La ragione di questo voto unanime e convinto, che spiega la stessa presentazione della mozione, risiede nella volontà di riaffermare, in maniera chiara ed indiscutibile, il sostegno dell'attuale maggioranza parlamentare alle nostre Forze armate, che svolgono quotidianamente un ruolo fondamentale a tutela degli interessi nazionali e di valori essenziali, quali la pace e la democrazia. È grazie al loro contributo che l'Italia gode oggi di un significativo prestigio internazionale e di un apprezzamento unanime nell'ambito di tutti i consessi mondiali. Non ho poco fa parlato a caso di volontà di riaffermare il sostegno del Popolo della Libertà ai militari di ogni Forza armata: perché, è bene ricordarlo, il nostro appoggio non è mai stato un elemento episodico ed accidentale, magari condizionato da ragioni di mera opportunità politica contingente. Il nostro sostegno alle Forze armate ed ai valori che le stesse rappresentano fa parte, per così dire, del nostro DNA. Fa parte della nostra visione politica, oggi come ieri, come sempre: sia quando siamo stati all'opposizione, sia oggi al Governo. Pertanto, dobbiamo e vogliamo respingere con forza l'idea secondo cui l'azione politica dell'attuale e del precedente Governo di centrodestra sia stata e sia tuttora diretta ad apportare tagli indiscriminati al bilancio della difesa e che tutto ciò possa essere considerato segnale di una scarsa attenzione per le esigenze delle Forze armate o, peggio, di una volontà di ridimensionamento della capacità operativa delle stesse. La crisi economica che ha colpito duramente tutte le economie mondiali negli ultimi mesi ha costretto - e non poteva essere altrimenti - il Governo italiano e la maggioranza che lo sostiene ad una politica di razionalizzazione delle risorse finanziarie pubbliche, pubbliche, politica che ha riguardato tutti gli stati di previsione del bilancio dello Stato. Questa tempestiva e decisa azione ha permesso al nostro Paese di affrontare al meglio l'attuale difficile situazione economica mondiale, come peraltro recentemente riconosciuto da autorevoli osservatori internazionali. A fronte di questa indispensabile - ed inevitabile - azione a garanzia dei nostri conti pubblici, sono però necessarie delle precisazioni. In primo luogo, è bene ricordarlo, in Italia la spesa pubblica relativa alla "funzione difesa", in percentuale sul prodotto interno lordo nazionale, negli ultimi anni è stata sostanzialmente stabile. A questa considerazione, che si potrebbe dire di macro-sistema, si devono aggiungere alcuni recentissimi eventi. Infatti, il decreto-legge anticrisi emanato pochi giorni fa dal Governo, ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, all'articolo 24 prevede il rifinanziamento delle missioni internazionali per il 2009 per una quota pari a 510 milioni di euro. Queste risorse finanziarie "fresche" vanno ad aggiungersi ai circa 800 milioni di euro già stanziati a febbraio con la conversione del decreto-legge di proroga delle missioni internazionali. Ciò comporta che, per l'anno 2009, questa maggioranza e questo Governo hanno già autorizzato per le missioni dei nostri soldati all'estero una spesa di circa 1,3 miliardi ben superiore al limite di un miliardo previsto per quest'anno dalla legge finanziaria 2007 del Governo Prodi. Allo stesso modo il collega Amato ha richiamato altre angolazioni analitiche da noi apprezzate. Questa rilevante quantità di risorse finanziarie permetterà di soddisfare integralmente le spese delle missioni all'estero, evitando così di dover utilizzare, a copertura delle stesse, disponibilità ulteriori provenienti dallo stato di previsione del Ministero della difesa. Inoltre, vorrei ricordare che lo stesso decreto-legge anticrisi ha stanziato altri 27,7 milioni di euro per l'anno in corso e 39,5 milioni di euro per l'anno 2010 per la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio. Dunque, nuove e rilevanti risorse finanziarie, cui si affianca una specifica azione finalizzata, non a ridimensionare, ma ad incrementare le capacità operative delle nostre Forze armate. Prova ne è la recente approvazione parlamentare di alcuni rilevantissimi programmi di investimenti pluriennali, finalizzati a mantenere sempre all'avanguardia il livello tecnologico della nostra Difesa. Onorevoli colleghi, la mozione che con forza sosteniamo ha un altro fondamentale obiettivo: garantire il sostegno del Parlamento italiano al processo in corso di ridefinizione del sistema complessivo di difesa e sicurezza nazionale. La fine della Guerra fredda e la caduta del Muro di Berlino, di cui proprio quest'anno ricorre il ventennale, hanno modificato indelebilmente il ruolo del nostro Paese - e quello delle sue Forze armate - nel contesto strategico internazionale. Si è assistito ad una sostanziale diminuzione della presenza in Europa e nel Mediterraneo di forze militari ostili, in grado di portare nel medio termine minacce dirette al territorio nazionale. Nello stesso tempo, da un lato, si sono moltiplicate in varie zone del mondo (Medio Oriente, Afghanistan, Iraq, Iran, Somalia), le crisi regionali, talune potenzialmente capaci di determinare significativi effetti sulla situazione geostrategica mondiale. Dall'altro, è emerso sulla scena mondiale il fenomeno del terrorismo internazionale globalizzato di matrice islamica, concretamente in grado - come si è potuto negli anni trascorsi tristemente accertare - di elevare l'entità del pericolo a livelli in passato inimmaginabili. Nuove ed impegnative sfide, alle quali l'Italia e le sue Forze armate hanno risposto con grande coraggio, senso del dovere, professionalità e capacità operative. Credo sia doveroso ricordare che oggi il nostro Paese è impegnato attivamente in più di 30 missioni internazionali con quasi 9.000 tra soldati, marinai, avieri, carabinieri e finanzieri. rilevante, che eleva l'Italia tra i primi Paesi al mondo negli interventi di pace ed a sostegno della democrazia e della legalità internazionale. Con questa mozione, quindi, vogliamo esprimere l'appoggio del Parlamento proprio a questo difficile ma inevitabile processo di cambiamento delle nostre Forze finalizzato a reagire nel modo più appropriato e con quella professionalità che le ha sempre contraddistinte alle nuove difficili imprese che il nostro Paese deve e dovrà affrontare nei prossimi anni. Esprimo, infine, un ringraziamento al Governo, al Ministro della difesa e a tutti coloro che operano in questo settore. Si tratta di far sì che le Forze armate possano continuare a disporre in futuro delle capacità operative necessarie per corrispondere adeguatamente alle esigenze di difesa dello Stato, assicurando, nell'ambito del sistema internazionale di sicurezza, un contributo coerente con il ruolo del nostro Paese, chiamato da domani ad ospitare, nella veste di presidente di turno, il *summit* del G8

e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Colleghi, per comunicare i risultati della Conferenza dei Capigruppo sul calendario dei lavori, sospendo la seduta

la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi pomeriggio, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 23 luglio. Domani mattina sarà innanzitutto esaminato il decreto-legge in materia di contrasto alla pirateria. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 20 di questa sera. Seguirà, sempre nella giornata di domani - se possibile fin dalla seduta antimeridiana - la discussione del disegno di legge collegato in materia di internazionalizzazione imprese ed energia, che si concluderà entro la mattina di giovedì 9 luglio. Per il voto finale di questo provvedimento è richiesta la presenza del numero legale. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro un'ora dalla conclusione dei lavori della Commissione competente. La prossima settimana, l'Assemblea si riunirà nella seduta pomeridiana di martedì 14 luglio per la discussione di mozioni sul caporale israeliano Gilad Shalit e sulla minoranza di lingua italiana in Croazia. Il resto della settimana sarà riservato ai lavori delle Commissioni, con particolare riguardo all'esame del DPEF e dei disegni di legge di rendiconto e assestamento del bilancio dello Stato. Nella seduta antimeridiana di martedì 21 luglio si svolgeranno le discussioni generali su mozioni in materia di sicurezza del trasporto ferroviario, G8 e promozione dell'energia solare. I tempi saranno ripartiti in modo da consentire la conclusione delle tre discussioni generali entro le ore 14. Le dichiarazioni di voto e le votazioni avranno luogo nel pomeriggio. Nella rimanente parte della seduta pomeridiana di martedì 21 luglio saranno esaminati documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che, ove non conclusi, potranno eventualmente proseguire dopo il voto dei documenti finanziari. Nella seduta antimeridiana di mercoledì 22 luglio sarà discussa una questione concernente autorizzazione a procedere per reati ministeriali. Le iscrizioni a parlare in discussione generale dovranno pervenire entro le ore 19 di martedì 21 luglio. Come previsto dall'articolo 135-*bis*, comma 8-*bis*, del Regolamento, la questione sarà posta ai voti con scrutinio nominale elettronico entro la fine della seduta antimeridiana. Successivamente, anche nel corso della seduta pomeridiana dello stesso giorno, i senatori che non abbiano partecipato alla votazione potranno dichiarare il proprio voto ai senatori Segretari fino alle ore 19. Nella stessa seduta pomeridiana di mercoledì 22 luglio inizierà la discussione del Documento di programmazione economico-finanziaria che si concluderà entro la seduta antimeridiana di giovedì 23. Nel corso della stessa settimana saranno anche esaminati i disegni di legge di rendiconto e assestamento del bilancio dello Stato. Ripartizione dei tempi e termini per la presentazione di proposte di risoluzione e di emendamenti ai predetti documenti finanziari saranno definiti dalla prossima Conferenza dei Capigruppo. Nella seduta pomeridiana di giovedì 23 luglio, alle ore 16, avranno luogo interrogazioni a risposta immediata con trasmissione diretta televisiva della durata di un'ora.

I chicchi di grandine hanno flagellato i vigneti in modo inaudito. Al momento si lavora per fare le prime stime dei danni e sicuramente si cercherà di intervenire anche *in loco* tramite la Giunta provinciale.

a cui il Comune di Milano lo scorso anno aveva affidato una parte di un lotto di appalto per servizi di vigilanza nei quartieri e persino sui convogli della metropolitana.

Tutti hanno dato segni di grande stupore e di assoluta sorpresa

Grazie, Presidente. spostando l'attenzione da Milano a Napoli, da un Comune ad una Regione importante qual è la Campania. Penso che, come nel caso della collega, il fatto che sia diventata definitivamente legge la normativa sulla sicurezza renda più facile la risposta ai nostri atti di sindacato ispettivo. Personalmente, insieme ad altri colleghi, se non proprio nel 2008 settimane prima dell'approvazione in Senato della normativa di cui si è parlato, avevo segnalato al Presidente del Consiglio, al Ministro dell'interno e al Ministro per gli affari regionali quanto avvenuto con ampia disponibilità di risorse, perché siamo su cifre assai più alte di quelle richiamate dalla collega per il comune di Milano. Trattasi, non già di ex poliziotti, ma di ex detenuti. La Regione Campania ha riservato 426 posti di volontario per la sicurezza turistica alla cooperativa degli ex detenuti. Dico questo con tutta la sensibilità che si deve alla condizione di queste persone, ma tenendo ben presente, come insieme ad altri colleghi segnalavamo in questo documentato atto di sindacato ispettivo, che quella della regione Campania è una scelta di buonismo e, nello stesso tempo, di cinismo. Non è ammissibile